lettura della lettera che il Presidente della Corte costituzionale ha inviato al Presidente del Senato: «Roma, 4 maggio 2007 Illustre Presidente, Le comunico che in data odierna la Corte, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale, ha accettato le dimissioni

Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 24 aprile 2007, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate

riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 maggio. Anzitutto l'ordine del giorno di questa seduta è integrato con un'informativa del Vice Presidente del Consiglio dei ministri - che interverrà alle ore 17,30 sulle dichiarazioni attribuite a componenti del Governo in merito al giudizio di ammissibilità del *referendum* elettorale da parte della Corte costituzionale. Nel successivo dibattito, per il quale non sono previste votazioni, potranno intervenire i Gruppi per 10 minuti ciascuno (15 minuti al Gruppo Misto). Successivamente la seduta sarà tolta. Saranno pertanto posti all'ordine del giorno di domani i disegni di legge già previsti per oggi: delega diritti televisivi calcio, rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione e due ratifiche di accordi internazionali; nonché le votazioni in materia di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali (queste ultime, a scrutinio elettronico, avranno luogo intorno alle ore 11,30-12, con successiva possibilità di esprimere il proprio voto palese ai senatori Segretari sino alle ore 19). Il calendario della corrente settimana comprende inoltre l'esame del disegno di legge per l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali. Per la prossima settimana il calendario prevede, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge sul ripiano della spesa sanitaria, se modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, nonché la sola discussione generale dei disegni di legge recanti modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 16 maggio si svolgerà la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Resta confermato che nella settimana successiva, in vista delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio, l'Assemblea non terrà seduta. Potranno invece convocarsi le Commissioni in relazione ai rispettivi calendari dei lavori. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa elettorale, sarà data priorità al disegno di legge recante delega al Governo sulla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

prima di dare la parola al vice presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Francesco Rutelli, che ringrazio per la sollecitudine con cui ha accettato l'invito a riferire al Senato,

giorno reca: «Informativa del Vice presidente del Consiglio dei ministri sulle dichiarazioni attribuite a componenti del Governo in merito al giudizio di ammissibilità del *referendum* elettorale da parte della Corte costituzionale». Ha facoltà di parlare il vice presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Rutelli.

a nome del Governo, intendo offrire, con la massima lealtà e con pieno spirito di collaborazione, ogni utile elemento informativo per la valutazione del Senato della Repubblica. È con questo atteggiamento di massima apertura che devo però sottolineare che proprio la posizione di indipendenza e di assoluta autonomia, che spetta istituzionalmente alla Corte costituzionale, deve definire rigorosamente il contenuto dell'intervento del Governo nell'ambito della presente discussione parlamentare. Pertanto, il mio discorso si incentra principalmente sull'obiettiva ricostruzione della vicenda all'esame del Senato, per poi riassumere, in modo essenziale e mi auguro puntuale, la posizione espressa in merito dal Governo, per la parte in cui esso è stato in qualche modo (e del tutto impropriamente, a mio giudizio) chiamato in causa. Il Governo è pienamente consapevole della circostanza che, in linea generale, le dimissioni di un giudice costituzionale, prima della scadenza naturale del mandato, costituiscano un fatto inusuale e serio. Esse suscitano l'attenzione dell'opinione pubblica e richiamano quella delle istituzioni, tanto più per la riservatezza che contrassegna tradizionalmente lo svolgimento dei compiti della Suprema Corte. Al riguardo, va sottolineato che, in precedenza, le dimissioni anticipate di un giudice costituzionale si sono verificate solo in due occasioni. La consapevolezza del possibile rilievo delle dimissioni diventa ancor più evidente ed acuta quando, all'origine dell'atto, il giudice dimissionario indica, espressamente e pubblicamente, il paventato rischio di una limitazione dell'indipendenza della Corte costituzionale determinata, a suo dire, dalle dichiarazioni rese, secondo alcuni organi di stampa - seppure si siano registrate successive smentite degli interessati - da alcuni Ministri e da un Sottosegretario in carica nell'attuale Governo. Per queste ragioni, il Governo, restando accuratamente nei confini delle proprie attribuzioni costituzionali, intende riaffermare con chiarezza, in questa sede (come ha già fatto, tempestivamente, in altri contesti istituzionali ed attraverso i propri comunicati ufficiali), posizione sull'episodio. Ecco la semplice descrizione cronologica dei fatti, che, a mio avviso, conferma l'assoluto rispetto per il ruolo della Corte costituzionale, quale istituzione di garanzia suprema del diritto e dell'ordinamento costituzionale. Il 30 aprile di quest'anno, il professor Romano Vaccarella rassegna le dimissioni dalla Corte, dopo averle anticipate verbalmente sin dal 28 aprile, con comunicazione inviata al Presidente ed al Vice presidente della Corte. L'atto viene motivato richiamando espressamente una notizia di stampa, secondo la quale alcuni esponenti dell'attuale Governo avrebbero svolto delle dichiarazioni, in materia di ammissibilità del *referendum* elettorale, giudicate - cito - «offensive della dignità e dell'indipendenza della Corte stessa». Il 29 aprile il presidente del Consiglio, onorevole Romano Prodi, esprimendo il convincimento dell'intero Governo, aveva riaffermato con chiarezza l'indiscussa necessità di rispettare costantemente la divisione dei compiti attribuiti alle massime istituzioni: un riconoscimento del ruolo di autonomia sostenuto, "naturalmente" anche con specifico riferimento ai compiti riguardanti il giudizio (sia pure futuro ed eventuale) sulla ammissibilità dei *referendum* elettorali. Questa attestazione di piena e, vorrei dire, ovvia conferma del rispetto del Governo per la Corte, i suoi giudici e le sue funzioni, viene ribadita dal Presidente del Consiglio, il giorno 30 aprile, anche di fronte alla stampa e poi ulteriormente ripetuta in una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio, secondo la quale - cito - «il Governo è pienamente consapevole della necessità di non interferire né direttamente né indirettamente nel lavoro della Corte costituzionale, verso la quale nutre il dovuto e totale rispetto». Il 30 aprile, il Quirinale dirama un comunicato stampa del seguente tenore: «Il Presidente della Repubblica ha ricevuto dal Presidente della Corte costituzionale comunicazione telefonica della lettera di dimissioni da Giudice Costituzionale del Professor Romano Vaccarella e delle sue motivazioni. In proposito, nel corso della conversazione, il Presidente della Repubblica ha ricordato i suoi precedenti interventi sulla necessità dell'assoluto rispetto da ogni parte dell'alta funzione di garanzia della Corte, chiamata ad esercitare in piena autonomia tutte le competenze attribuitele dalla Costituzione». Il 2 maggio, la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, delibera, all'unanimità, di respingere le dimissioni del giudice Vaccarella. Questo il testo della pronuncia: «La Corte costituzionale, considerato che alcuni quotidiani il 25 ed il 26 aprile u.s. hanno attribuito ad esponenti del Governo dichiarazioni relative alla posizione della Corte in tema di ammissibilità di *referendum* su leggi elettorali; e che a seguito di tali dichiarazioni non smentite, il giudice costituzionale, professor Romano Vaccarella, per protesta, il 30 aprile rassegnato le dimissioni dalla Corte; considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affermato il 29 ed il 30 aprile la necessità del rispetto del ruolo istituzionale della Corte e della totale sua indipendenza ed autonomia, negate dalle dichiarazioni riportate dagli organi di stampa, il cui contenuto deve quindi considerarsi nella sostanza disapprovato dal Governo; considerato inoltre che il Presidente della Repubblica ha ricordato i suoi precedenti interventi sulla necessità dell'assoluto rispetto da ogni parte dovuto all'alta funzione di garanzia della Corte stessa; e che anche i Presidenti del Senato e della Camera hanno sottolineato l'indipendenza e l'autonomia della Corte; considerato che occorre ribadire la necessità che esponenti di altre Istituzioni evitino comportamenti denigratori della Corte, come le dichiarazioni suddette, e rispettino il suo ruolo di garanzia costituzionale,

irrevocabilmente, le proprie dimissioni dalla Corte costituzionale. Lo stesso giorno la Corte delibera la presa d'atto delle dimissioni. Questo il testo infine della pronuncia: «la Corte costituzionale, preso atto che, con nota in data odierna diretta al Presidente, il giudice costituzionale professor Vaccarella ha confermato in modo irrevocabile le sue dimissioni dalla carica, richiamate le considerazioni di cui alla delibera del due maggio e riaffermato che la propria indipendenza è garantita istituzionalmente dalla collegialità del suo operare, delibera all'unanimità di accettare le dimissioni del giudice costituzionale professor Romano Vaccarella». Essendo questa, oggettivamente, colleghi senatori, la successione dei fatti che hanno condotto alle dimissioni del giudice Vaccarella, il Governo non intende e non può svolgere commenti o valutazioni sulla personale decisione finale di dimissioni assunta dal professor Vaccarella. L'indipendenza e l'autonomia della Corte e dei suoi giudici impediscono qualsiasi interferenza sulle scelte che conducono alla nomina, in questo caso nomina parlamentare, dei componenti della Corte costituzionale e, a maggior ragione, non spetta al Governo prendere posizione sulle autonome determinazioni di singoli giudici di lasciare l'incarico prima del termine di scadenza. Sarebbe del resto superfluo, signor Presidente, anche in questo contesto, ribadire il senso di altissima considerazione per i profili professionali, culturali, istituzionali che caratterizzano da sempre la storia della Corte costituzionale, sviluppatasi ormai in più di mezzo secolo di vita della Repubblica. Non sono mancate, a più riprese, espressioni di giudizio su decisioni della Corte, anche di tenore critico. Esse, va ricordato, sono legittime come in tutti i casi in cui ci si confronta con l'esercizio della giurisdizione. E si sono registrate, in passato, anche prese di posizione preventive da settori sociali, politici, parlamentari alla vigilia di pronunzie della suprema Corte. Ciò non ha mai portato, tuttavia, a far ritenere che le successive decisioni della Corte siano state condizionate, o in alcun modo influenzate, da tali prese di posizione. dell'autorevole senatore Manzella che, citando il Manzoni e il suo celebre: «la sventurata rispose», chiarisce a suo modo che la Corte costituzionale non è «sventurata» e, in principio, non risponde. Mi limito a richiamare, a questo proposito, il passaggio della delibera del due maggio della Corte costituzionale in cui si riconosce la presa di posizione del Governo che contrasta e disapprova ogni condotta diretta a minare l'autonomia e l'indipendenza della Corte stessa. Quindi, proprio questa asettica descrizione dei fatti conferma che, per il Governo, così come la divisione dei poteri tra le istituzioni della Repubblica costituisce riferimento invalicabile degli organi costituzionali. In nessun modo si deve confondere questo assunto con l'espressione di valutazioni e di giudizi che, in una democrazia, certamente è legittimo riscontrare, anche se non sempre,

invalicabile solo attraverso dichiarazioni o affermazioni di principio, che pure rispecchiano le profonde convinzioni della nostra idea di democrazia costituzionale, la nostra incondizionata adesione ai principi dello Stato di diritto, ma si concretizza nella dinamica di svolgimento delle funzioni attribuite ai massimi organi costituzionali. Noi vorremmo, colleghi, e concludo, che la stessa posizione di rispetto della Corte costituzionale e di lealtà verso le istituzioni repubblicane fosse mantenuta sempre e da tutti, anche dagli esponenti di forze politiche, i quali spesso, anche in un recente passato, rivolgendosi alla Corte costituzionale, hanno utilizzato toni assolutamente inaccettabili. Credo che la conclusione di questa vicenda, sancita dalla Corte stessa, che, signor Presidente, all'unanimità ha riaffermato sia la propria indipendenza, sia la garanzia assicurata dalla propria collegialità, debba consigliare tutti, membri del Parlamento e del Governo, altri titolari di cariche istituzionali, esponenti della politica, di concludere ogni polemica e anche di abbassare i toni, nell'interesse del sereno esercizio dei compiti che la Costituzione affida in modo libero e responsabile a tutte le istituzioni repubblicane. *(Applausi

*(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il dibattito odierno riguarda un caso che conta soltanto due precedenti nella storia della Repubblica italiana, un caso scandito da una strana tempistica coincidente con la tanto dibattuta questione del *referendum* Guzzetta-Segni sulla legge elettorale. un caso riguardante un singolo giudice e le sue interlocuzioni sulla carta stampata con esponenti di Governo, interlocuzioni caricate dei più svariati significati. Dalla specifica vicenda sono affiorate le più composite problematiche di ordine politico-istituzionale, che, certamente, in questi brevi minuti di dibattito parlamentare, non potranno essere affrontate con pretese di esaustività. Si passa da questioni inerenti le dinamiche interne del supremo organismo giurisdizionale, ai rapporti (o, come si preferisce definirli, intromissioni, pressioni, ingerenze) tra questo organismo e gli altri protagonisti della vita politica, al ruolo della Corte nel giudizio di ammissibilità dei dei *referendum* concernenti la materia elettorale. Quanto alla stretta dinamica delle dimissioni e cioè la presentazione di queste, il loro rigetto da parte della Corte, gli innumerevoli inviti al ritiro, la riconferma delle stesse da parte del giudice Vaccarella, che questi abbia effettivamente mostrato credibilità e serietà. Il suo convincimento circa l'ammissibilità dei quesiti referendari, infatti, come ben ha fatto notare il ministro della giustizia Mastella, non sarebbe stato certamente immune da valutazioni travalicanti il merito giuridico. il merito giuridico. Quanto, invece, alla propugnata difesa del suo ruolo fino all'estrema conseguenza delle dimissioni, penso che il giudice non abbia forse attribuito la giusta misura a due considerazioni fondamentali: innanzi tutto, che la intercomunicabilità tra organi dello Stato non è sinonimo di interferenza. È infatti inconcepibile pensare che le istituzioni democratiche siano monadi prive di qualsiasi possibilità di interlocuzione, che protagonisti della vita pubblica non possano esprimere riflessioni libere ed autonome. L'ammissibilità del *referendum* sulla legge elettorale è inevitabilmente oggetto di riflessione politica e di disamina da parte di costituzionalisti che non si sono certo tirati indietro dal manifestare i propri convincimenti, tanto a sfavore quanto a sostegno, sul punto. Si pensi, ad esempio, da una parte, alle opinioni del professor Lippolis, che riflette, addirittura, circa la possibile evoluzione della Corte di esprimere un giudizio di costituzionalità anticipato sulla normativa di risulta del *referendum*, che in questo caso produrrebbe un risultato di macroscopica incostituzionalità. Si pensi, d'altra parte, alle opinioni del professor Morrone a sostegno della chiarezza, della non manipolatività o dell'autoapplicatività del quesito referendario. Dunque, dovrebbe essere messo il bavaglio ai costituzionalisti o ai politici? La risposta è, ovviamente, scontata. La seconda riflessione attiene invece alla Corte costituzionale, quale istituto collegiale: la forza e l'autonomia dell'organismo dipendono proprio da ciò. Vorrei concludere riportando testualmente le parole del professor Onida, presidente emerito della Corte, apparse su «Il Sole 24 ORE» il 3 maggio scorso: «Sulle questioni controverse, i singoli giudici possono volta a volta trovarsi a comporre la maggioranza della Corte o restare in minoranza, ma ciò non è mai frutto meccanico di "schieramenti" presenti al suo interno e, tanto meno, il riflesso di "schieramenti" esterni, bensì il risultato, talvolta imprevedibile, di una dialettica interna che si apre di volta in volta su ciascun argomento». *(Applausi

aperto un dibattito nel Paese e in Parlamento molto importante sul piano politico. La risposta del vice *premier* Rutelli non poteva che essere quella che ci è stata fornita,

sostenere che il Governo nulla ha fatto nei confronti dei giudici costituzionali per far rendere inammissibili i quesiti referendari.

anche recentemente, un ex Presidente della Corte costituzionale lo ha ammesso con assoluta chiarezza). Non dobbiamo nasconderci, quindi, dietro a un dito: su questo *referendum* si sta giocando una partita fondamentale per il sistema politico italiano. Soprattutto le forze politiche e i partiti piccoli e medio-piccoli si sentono profondamente

finirebbe questo sistema istituzionale partitico che non garantisce né governabilità né stabilità. Allora, è evidente che le forze politiche non devono interrogarsi su come escogitare sotterfugi o esercitare pressioni sulla Corte costituzionale per bloccare il *referendum*, ma devono sedersi attorno a un tavolo e ragionare su come, dopo 15 anni di questa cosiddetta Seconda Repubblica, si debba costruire un sistema elettorale istituzionale che, finalmente, consenta al nostro Paese di essere governato in modo diverso e serio. Tutti oggi, in in quest'Aula, in Italia, sono affascinati dall'esito delle ultime elezioni francesi, da questo chiarissimo e nuovo confronto tra destra e sinistra, tra centro-destra e centro-sinistra, tra uomini nuovi che finalmente abbandonano gli schemi ideologici

affrontata in modo assolutamente diverso. Io mi auguro intanto che il *referendum* venga dichiarato in qualche modo ammissibile e che, nei prossimi mesi, le forze politiche abbiano la capacità di fare un salto di qualità

Starà alle forze politiche, alla loro intelligenza e alla capacità di cogliere l'occasione offerta loro per aprire una fase nuova che, finalmente, dia all'Italia un sistema di alternanza veramente valido e in grado di farci fuoriuscire dalla tragica situazione nella quale siamo caduti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice presidente del Consiglio, il Gruppo Per le Autonomie ha ha apprezzato molto l'equilibrio del suo intervento e anche il senso delle istituzioni che lo ha animato. Si tratta, indubbiamente, di un passaggio molto delicato per il nostro sistema democratico perché, come il il ministro Rutelli ha ricordato, è un evento molto raro nella storia della Repubblica. Le dimissioni di un giudice costituzionale sono un fatto grave, questo caso per le ragioni che lo hanno motivato, cioè la convinzione del giudice Vaccarella che la Corte non sia nelle condizioni di giudicare serenamente dell'ammissibilità del *referendum* sul quale si stanno raccogliendo

Corte, l'opinione pubblica ha il diritto di conoscere quali sono le ragioni precise di tali accuse. È difficile pensare che la Corte possa essere violata nella sua autonomia da dichiarazioni di questo o quel Ministro, di questo o quel Sottosegretario. Dichiarazioni che, peraltro, personalmente non condivido (come è noto, faccio parte del Comitato promotore del *referendum*), anche se credo sia difficile giustificare l'esistenza di una limitazione all'autonomia della Corte costituzionale motivata sulla base di qualche intervista giornalistica. È infatti

Nessuna Corte suprema, nessuna Corte costituzionale, nel momento in cui valuta la costituzionalità di una norma o, come in questo caso, l'ammissibilità di un *referendum*, può prescindere del tutto dal contesto politico e storico nel quale un Paese si trova. Ce lo insegna, del resto, l'esperienza del Paese che tutti consideriamo la patria della democrazia contemporanea, gli Stati Uniti d'America: tutti sanno che la Corte suprema ha un suo indirizzo politico e che l'elezione di questo o di quel giudice della Corte può cambiare l'indirizzo politico in un punto essenziale del funzionamento di un sistema democratico complesso e delicato come quello degli Stati Uniti d'America. E tuttavia, un conto è il giudizio politico che la Corte, ovviamente a partire dal suo punto di vista, che è quello della corrispondenza tra la decisione che deve assumere e la Costituzione, formula in assoluta autonomia, altra cosa sarebbe un giudizio politico che dovesse invece essere formulato sulla base di pressioni indebite e di interferenze operate da altri poteri. Questo sarebbe un fatto molto grave, che metterebbe a repentaglio la credibilità delle nostre istituzioni e l'accessibilità, nel caso specifico, da parte dei cittadini, ad uno strumento essenziale di democrazia, qual è il *referendum*. tuttavia, noi confermiamo, signor Presidente, la fiducia piena nella capacità della Corte costituzionale di formulare il giudizio di ammissibilità, in questo, come in tutti gli altri casi, in modo assolutamente autonomo e sovrano, avendo presente soltanto, così dire, da un lato, la lettera e lo spirito della Carta costituzionale e, dall'altro, la valutazione di coscienza di ciascun giudice e della Corte nella sua collegialità. Confermiamo la piena fiducia alla Corte costituzionale e al suo presidente Franco Bile, magistrato di nota e specchiata onestà e consolidata indipendenza dalla politica, e siamo convinti che in una società libera e democratica, qual l'Italia è, la Corte possieda tutti gli strumenti per far valere la sua piena indipendenza e la sua piena autonomia. In un Paese come il nostro, non si è autonomi e indipendenti solo se si accetta di non esserlo: se si vuole esserlo, lo si è, perché la Costituzione è a presidio delle libertà di tutti e dell'autonomia di ciascuna istituzione.

gravi di intimidazione nei confronti di esponenti del movimento referendario che stavano esercitando un preciso diritto costituzionale: erano, in quel momento, una istituzione della Repubblica all'opera. Questi episodi non devono essere in alcun modo minimizzati e credo che da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni (quindi, il Governo per la sua parte, ed abbiamo apprezzato le parole

Come Gruppo IU-Verdi-Com, abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà al dibattito, perché l'abbiamo considerato inutile e per alcuni versi anche pericoloso,

Tutto sembrerebbe nascere da un retroscena, pubblicato sui giornali, in cui venivano riportate opinioni di personaggi politici influenti sull'ammissibilità o meno del *referendum* (di cui personalmente penso tutto il peggio possibile). Ma da quando esprimere le proprie opinioni - Ministri o no che si sia - significa fare pressioni illecite sulla Corte o compiere un atto illecito? È una cosa del tutto legittima: le opinioni, da chiunque vengano, anche da Ministri, Sottosegretari o politici, non sono sindacabili, mai. La seconda ragione mi sembra più delicata. La Corte costituzionale è, nella divisione dei poteri, un organismo di garanzia; è perciò autonomo e la sua autonomia va rigorosamente rispettata. Proprio per questo, però, onorevoli senatori, è all'interno della Corte e in nessun altro luogo istituzionale - a mio avviso - che vanno discusse eventuali dimissioni. Questo dibattito io lo avverto come una sorta di interferenza e inoltre - voglio dirlo con grande franchezza - le dimissioni del professor Vaccarella hanno qualcosa di strumentale, persino di poco corretto: non sono state indirizzate solo al Presidente della Consulta, come il professor Vaccarella avrebbe dovuto fare, ma anche ad altri organi politici ed istituzionali, rompendo il tradizionale riserbo della Corte, che non è un fatto di buone maniere ma di opportunità istituzionale, ed alimentando così le polemiche giornalistiche. Il professor Vaccarella è evidentemente un uomo impulsivo, io non lo conosco e non mi azzardo a dare di lui alcun giudizio. Mi permetto però di ricordare all'opposizione - anche se può sembrare sgradevole, ma non è questo - le parole di Filippo Mancuso il giorno della sua elezione: «Sono riusciti a portare lo studio Previti alla Corte costituzionale». Non mi risultano, in quell'occasione, reazioni del professor Vaccarella. In realtà, credo si stia facendo molto rumore per nulla e in qualche misura quest'Aula, al di là del dibattito abbastanza agitato in Conferenza dei Capigruppo, sembra dimostrarlo. Invece Invece di discutere le dimissioni del giudice, cosa assai delicata, bisogna eleggerne velocemente il sostituto. Non credo che si possa accusare il centro-sinistra di aver mai mancato di rispetto alla Corte costituzionale: per storia, per tradizione, per formazione abbiamo un forte rispetto delle istituzioni. Altri lo hanno fatto, però, e in anni anche recenti. Si può mancare di rispetto in vari modi, non in uno solo: individuando la Corte, per esempio, come Berlusconi ha più volte fatto, come un covo di comunisti, protestando per le sue sentenze o addirittura ignorandole. Penso a quando la Consulta dichiarò illegittima la legge Pecorella o quando, nel 1994, sentenziò l'incostituzionalità delle reti televisive concesse a Berlusconi; penso ai commenti, qualche volte ai limiti dell'insulto, quando dichiarò incostituzionale il lodo Schifani e l'ex Cirielli. Vorrei poi ricordare un episodio: un giorno l'onorevole Bossi accusò la Corte di avere bloccato il federalismo e di essere - disse - il nemico giurato delle Regioni; allora, la Corte se la prese, ci furono proteste, anche rimproveri, ma non fece nessun atto politico strumentale, come invece appare quello del professor Vaccarella. Allora, l'onorevole Ignazio La Russa difese Bossi dicendo (parole testuali): «Oltre che Ministro, è un *leader* politico e può tranquillamente esprimere le proprie opinioni». Sono d'accordo, è vero; in quell'occasione, aveva ragione l'onorevole La Russa. Anche i ministri Pecoraro e Chiti hanno espresso le loro opinioni, ma nell'opposizione ci deve essere stato un sussulto d'intolleranza che l'ha avuta vinta sulla ragione. Noi speriamo, signor Presidente, che questa storia finisca qui; che si elegga in fretta il sostituto del professor Vaccarella, che le istituzioni facciano il loro dovere senza sconfinamenti, come, per certi versi, è questo dibattito in Aula. E mi auguro che l'opinione pubblica non dia un giudizio troppo severo della politica, del suo parlare a se stessa. La gente vuole risposte concrete ai problemi della vita, onorevoli senatori, ai salari bassi, al lavoro precario; i problemi veri non sono certo le dimissioni del professor Vaccarella.

sul fatto che in un dibattito così importante la presenza del Vice presidente del Consiglio dei ministri è certamente significativa e autorevole. Tuttavia, attraverso lei, signor Presidente del Senato, vorrei invitare il Vice presidente del Consiglio dei ministri a prestare attenzione al dibattito perché se questa è diventata un'Aula all'interno della quale, fatto l'intervento scritto, il signor Vice presidente del Consiglio dei ministri poi riceve i *clientes* e ascolta

anziché stigmatizzare la denuncia del peccato, cercheremo di parlare del peccato e vedere se esso per caso c'è stato o meno. Io sono stato c'è stato o meno. Io sono stato attento quando parlava il Vice presidente del Consiglio e quindi cito testualmente le sue parole: «Per il Presidente del Consiglio la dimissione di un giudice costituzionale su un tema così devastante è un fatto inusuale e serio».

distratta o comunque quasi vuota. Questo, in qualche modo, forse giustifica anche l'atteggiamento del Vice presidente del Consiglio. Io invece credo che un tema del genere, che può e, secondo me, deve essere allargato al rapporto tra le varie istituzioni dello Stato, che a mio avviso - in questi anni è drogato e patologico, avrebbe meritato una platea e un interesse forse più vasto. Che cosa è accaduto? Uno dei fatti Uno dei fatti curiosi è che, con una preveggenza inusuale - questa sì - il presidente Prodi, addirittura il giorno prima delle dimissioni del professor Vaccarella, fatto un'affermazione che non poteva essere diversa. È chiaro che qualsiasi fariseo non può far altro che dichiarare che le istituzioni devono essere rispettate, che i poteri dello Stato devono devono essere indipendenti l'uno dall'altro e che vi sono alcuni organi di assoluta garanzia costituzionale. Cos'altro si potrebbe dire? Il problema è vedere poi, in pratica, cosa accade. Il professor Vaccarella - che conosco - è una persona seria, senatrice Palermi, e mi dispiace che lei abbia cercato d'infangarlo in questo modo,

in termini decisivi e problematici, è la seguente: la Corte riceve pressioni di questa natura da altri organi dello Stato? La Corte è permeabile politicamente? La Corte è connotata politicamente?

Fa parte della Corte costituzionale - e oggi ne è addirittura Vice presidente - un esimio giurista, che però è stato Ministro politico di un Governo Prodi: il professor Flick. dunque, non è stato un Ministro soltanto tecnico e quindi chiamato per le sue capacità di natura tecnica; no, è stato un Ministro politico. Questa è la prova provata che in questo momento esiste nella Corte costituzionale una persona che era schierata politicamente.

sono influenze di natura politica; allora, lei è d'accordo con me nell'avere questi dubbi e questi sospetti. Credo che il Senato dovrebbe porsi questi problemi e rispondere

avendolo vissuto nei cinque anni precedenti, quanto fosse difficile vincere il percorso a ostacoli che spesso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale hanno posto nel cammino dell'azione del Governo Berlusconi. Questo è un dato di fatto. hanno impedito di guidare il Paese in un certo modo. Questo è un tema sul quale dobbiamo interrogarci perché quando

che le affermazioni e le lacerazioni delle vesti che sono state compiute in Aula, dicendo: «Per carità, non bisogna nemmeno mettere in discussione l'imparzialità assoluta, costituzionale sia della Corte che del Presidente della Repubblica», siano poi vere. Cito il fatto, affinché non vi sia alcun dubbio al riguardo, che noi siamo tra i primi a non voler questo *referendum*. Quindi, le pressioni, che a noi risultano esserci state nei confronti dei giudici, potrebbero farci comodo dal punto di vista politico, però, è evidente che non possiamo far altro che respingere questi metodi. Spero che su questo il Senato sia unanime.

questo dibattito ha qualche aspetto di particolare rilevanza e di particolare delicatezza. A differenza di quanto é stato detto in quest'Aula, credo che sia un dibattito utile e non pericoloso.

istituzionale che si è posta, sgomberando il terreno da ciò che è l'apparenza. Nessuno chiede al Governo di dire cosa pensa dell'indipendenza della Corte costituzionale; nessuno pensa di chiedere agli esponenti politici di questo Parlamento di non esprimere opinioni sulle decisioni della Corte costituzionale; nessuno pensa pensa per un momento di chiedere alla Corte costituzionale di operare senza rendersi conto delle conseguenze politiche delle sue decisioni. Noi stiamo discutendo di un'altra cosa. Chiedo una cortesia: onestamente, il collega Rutelli ha ragione

Lo dico a tutela dell'onorevole Rutelli, perché lui è lì e non può impedire a nessuno di noi di avvicinarsi a lui; lui è attento e se diventa disattento è irresponsabilità nostra. Siccome questo dibattito la fortuna di avere il Vice presidente del Consiglio presente, che ha riferito su questa vicenda, è molto importante che il Vice presidente del Consiglio ci ascolti. Do per scontato che conosca la questione reale ed istituzionale al centro della nostra attenzione che, lo ripeto ancora una volta, non è la richiesta dell'opinione del Governo sull'indipendenza della Corte.

che la decisione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del *referendum*, qualora saranno raccolte le firme necessarie per poterlo indire, sarà una decisione decisiva per la vita del Governo. Questa è la questione. È una decisione che mai la Corte costituzionale italiana ha dovuto assumere dal 1956 ad oggi in riferimento alla sorte dell'esistenza del Governo. Questa è la questione istituzionale. È del tutto ovvio che, all'interno del Governo, vi sono forze politiche che hanno dichiarato espressamente non di avere un'opinione sulla Corte, ma che, qualora il *referendum* fosse dichiarato ammissibile, darebbero vita alla crisi di Governo. Non è un'opinione sulla Corte costituzionale; è un'opinione politica sulla maggioranza di Governo. Questa è la questione. Si può ritenere che il Governo, la cui sorte dipende anche dalla decisione della Corte costituzionale, possa rimanere indifferente rispetto a tale decisione? Questa è la questione che poniamo al Governo in carica, al Governo Prodi e al vice presidente Rutelli. Non vogliamo sapere cosa pensa dell'indipendenza della Corte, come se fossimo in un seminario di diritto costituzionale. Ritengo che il giudice Vaccarella avesse immaginato che il Presidente del Consiglio dovesse dire non che le opinioni di alcuni Ministri o Sottosegretari

non sono tali da modificare l'orientamento del Governo nei confronti della Corte costituzionale. Questo è mancato nelle parole del Presidente del Consiglio, non l'opinione sull'indipendenza della Corte, ma la irrilevanza della decisione della Corte ai fini dell'esistenza del Governo. Poteva Prodi dir questo? A mio giudizio no, perché Prodi è il primo a sapere che la sorte del suo Governo si gioca largamente in vista del *referendum*. E perché si tratta di una questione di ordine politico-istituzionale? Perché tutti diamo per scontato che il *referendum* in quanto tale modificherebbe radicalmente la natura dell'alleanza che regge il Governo, dando vita ad una possibilità astratta, non concreta (dipenderà poi dalla volontà delle forze politiche), che forze politiche oggi decisive per la vita del Governo non lo siano più in conseguenza di quel *referendum*. È evidente che questa è la ragione che potrebbe portare alla crisi di Governo. È in grado il Presidente del Consiglio di dire che è indifferente rispetto a questo fatto? Io non ritengo che sia in grado di dirlo. Lo posso dire perché sono tra quelli che, quando il Governo Prodi si presentò per la nuova fiducia qualche mese fa, dissero espressamente che è il Governo Prodi in quanto tale l'ostacolo alla riforma elettorale. Questa era l'opinione che era di parte politica, che confermo oggi come opinione costituzionale. Il Governo Prodi è composto da una maggioranza all'interno della quale vi sono alcune forze politiche i cui

Questo è un argomento di ordine costituzionale ed istituzionale al quale il Vice presidente del Consiglio non ha dato e, secondo me, non poteva dare risposta. Questa è la questione sulla quale il Presidente del Consiglio era stato chiamato ad esprimere un'opinione, non l'indipendenza della Corte. E quando il Presidente del Consiglio dice di chiedersi il motivo di queste dimissioni, avvalora la tesi in base alla quale c'è una questione costituzionale riguardo alla natura del Governo.

Quindi, la raccolta delle firme sarà già un fatto rilevante; e la decisione della Corte sarà un fatto decisivo. Do per scontato che, in vista di quella decisione, all'inizio di gennaio dell'anno venturo, si riaccenderà il dibattito sull'autonomia della Corte costituzionale.

la questione di Governo. Mai le due precedenti dimissioni avevano neanche lontanamente riguardato la sorte del Governo in carica: né le dimissioni di De Nicola nel 1956, né quelle di Ferrari circa 15-20 anni dopo. Siamo in presenza, per la prima volta, di una questione di Governo decisa,

della sua maggioranza. Questa è la ragione: non il *referendum*, sul quale Vaccarella ha detto che le opinioni rimangono integre, ma la mancata risposta del Governo su tale specifica Questo è il motivo per il quale mantengo l'opinione che l'attuale Governo non possa sopravvivere all'indizione del *referendum* e che, mai come in questo caso, la Corte costituzionale abbia un compito decisivo sulla vita dell'Esecutivo. Non è questione di autonomia della Corte, ma di rapporti costituzionali tra Governo e Corte costituzionale. Un'ultimissima considerazione

La formazione della Corte, poi - non sottovalutiamo questo fatto - vorrebbe tendere all'imprevedibilità dei comportamenti politici. Si prevede, infatti, che un terzo dei giudici sia di provenienza magistratuale, prevalentemente legata all'età;

farebbero bene a non occuparsi della vita in carica del Governo che sostengono.

autonomia è un bene di importanza troppo grande e troppo preziosa per le istituzioni, prima ancora che per le forze politiche,

affinché quest'autonomia non sia compromessa da nessuna istituzione e da nessuna posizione politica. Rispetto a questo, dobbiamo dobbiamo valutare se l'atto delle dimissioni del giudice Vaccarella e soprattutto - insisto sul soprattutto - il dibattito politico e il significato che sul piano politico si è voluto dare a questo atto

nel merito e nel modo. Nel merito, innanzitutto, considerando che la Corte potrebbe essere influenzata da dichiarazioni, riportate dalla stampa, di Ministri e di Sottosegretari, cioè di esponenti del Governo. Bene; qui è stato definito improprio dal ministro Rutelli; altri hanno parlato di atto sproporzionato,

nel Paese che può ritenere che la Corte sia influenzabile da dichiarazioni di alcuni Ministri, quali quelle che sono state riportate? Se poi il presidente Castelli ha altre informazioni che a me non risultano, ma a cui nemmeno il giudice Vaccarella ha fatto riferimento - ha parlato di pressioni, di telefonate, di rapporti - evitiamo di enfatizzare e di andare a caccia di sospetti e di cose che non stanno nemmeno nella ricostruzione dei fatti.

proprio quelle virgolettate di cui si parla implicano o potevano implicare implicitamente una intenzione, più o meno consapevole, consapevole, o la pretesa che la Corte potesse o dovesse attenersi a quelle valutazioni. valutazioni. Già solo prospettare questo, significa mettere seriamente in pericolo, nella sostanza e nel merito, l'autonomia di giudizio della Corte, perché non vi è dubbio che qualunque giudizio la Corte esprima, avrà delle implicazioni politiche. Come qualcuno prima di me ha già detto, un giudizio di costituzionalità è sempre anche un giudizio politico,

in particolare, tagliando e ritagliando - come richiede appunto il *referendum* abrogativo - una legge esistente, disegna un'altra legge elettorale;

posso ritenere in quest'Aula, in questa istituzione, che vi sia un problema di costituzionalità, di uso appropriato di quello che la Costituzione definisce per il *referendum*. Questo vuol dire che sto pregiudicando il giudizio di ammissibilità o non ammissibilità che la Corte esprime? Mi preoccupano un po' anche i termini con cui ha posto la questione il presidente D'Onofrio. Non vi è dubbio che il *referendum*

allora, dobbiamo sovraccaricare di questo significato ed addirittura tradurre in questione istituzionale la decisione della Corte? Inviterei tutte tutte le parti politiche a fare molta attenzione a non enfatizzare ed a non caricare di una funzione impropria il giudizio della Corte. Vengo al secondo aspetto, riguardante l'atto delle dimissioni del giudice

così preziosa e così importante in una posizione politica; la esponiamo alle strumentalizzazioni delle parti politiche e mi pare che, se in qualche modo l'atto improprio e sproporzionato del giudice Vaccarella è già andato in questa direzione, spetterebbe a noi non seguirlo. *(Applausi dai Gruppi

non succede molto spesso, anzi ben si può dire che non era mai accaduto prima d'ora, che il Governo fosse chiamato in una delle Camere così recita il nostro ordine del giorno di oggi - a riferire su «dichiarazioni attribuite a componenti del Governo in merito al giudizio di ammissibilità del *referendum* elettorale da parte della Corte costituzionale». Forse, invece, è altre volte successo, ma grazie al cielo, non certo di sovente, che il Senato, signor Presidente, sia stato chiamato a discutere di una vicenda che non è quella che è indicata nel suo ordine del giorno.

con il che nulla avrebbe oggi da riferire il Vice presidente del Consiglio. Non l'ha fatto Francesco Verderami, che è colui il quale, con l'articolo pubblicato il 26 aprile scorso sul «Corriere della Sera», ha di fatto posto l'argomento all'ordine del giorno di questa seduta. Non l'ha fatto, ovviamente e men che meno, il professor Vaccarella, il quale, letto come tutti l'articolo «incriminato» e ascoltato per quattro giorni, che per un galantuomo qual è lui immagino siano stati lunghi e dolorosi, stati lunghi e dolorosi, l'assordante silenzio del Presidente del Consiglio, l'assordante silenzio dei personaggi della politica chiamati in causa dall'articolo, del Governo nel suo complesso e dei *leader* del centro-sinistra, ha preso carta e penna e, in una solitudine che non gli invidio, ha comunicato al suo Presidente, al Presidente della Corte costituzionale, che lui non era affatto d'accordo, non già a sentire o a leggere dichiarazioni di «componenti del Governo in merito al giudizio di ammissibilità del *referendum*» ma, ben diversamente e con un grado assoluto di rilevantissima gravità, che nessuno dentro e fuori quest'Aula ha titolo di revocare in dubbio, a sentire o a leggere dichiarazioni non tanto attribuite, signor Presidente, quanto piuttosto non smentite o non sufficientemente e convincentemente smentite, del Ministro Guardasigilli, del Ministro dell'ambiente, finanche del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i rapporti con il Parlamento, su quanto la Corte costituzionale sarebbe stata accomodante nell'esprimere un giudizio di inammissibilità che negasse in radice il diritto, la potestà dei cittadini di direttamente esprimersi su un argomento delicatissimo quale è quello della scelta del percorso da cui prende avvio la modalità con cui il Paese sarà governato: coerente con quella che tipizza le grandi democrazie dell'Occidente e non solo, ovvero vivacchiante come ancora oggi è nel «gioco degli ostaggi» che il sistema di microframmentazione consente. Perché è di questo, signor Presidente, che oggi in verità qui si discute; perché è di questo, signor Presidente, che oggi, in verità, il Vice presidente del Consiglio ha riferito al Parlamento. Il professor Vaccarella, il giudice costituzionale Vaccarella non ha certo bisogno di interpreti o di difensori, di fiducia o d'ufficio, né certo io avrei la presunzione di potermi candidare all'improbabile compito; né di interpreti o difensori ha bisogno la Corte costituzionale. Il professor Vaccarella, nel nitidamente sollevare la questione, nella sobrietà delle motivazioni portate alla propria decisione, non ha minimamente posto in dubbio che i giudizi della Corte costituzionale, di ammissibilità o meno di un quesito referendario piuttosto che in qualsiasi altra materia, possano essere oggetto di dibattito: giuridico, sociale, politico, culturale e in quanti altri contesti si voglia. Ci mancherebbe altro che proprio l'istituzione che lo Stato si è posto a custode permanente della conformità delle sue leggi al proprio assetto costituzionale e quindi a massimo presidio della scelta democratica a suo tempo stabilita come suo cardine,

Non è questo ciò di cui oggi si discute; non è questo ciò che ha indotto il giudice Vaccarella a rassegnare e a confermare le proprie dimissioni. Ciò che ha indotto il professor Vaccarella a comunicare e a confermare le proprie dimissioni nemmeno è la rozza e incauta esternazione di chi pure ha rilevanti e centrali responsabilità di Governo (mi riferisco, in particolare, al Ministro Guardasigilli e, ancor di più, al sottosegretario Naccarato, che ha la delicatissima funzione di cerniera fra poteri dello Stato), ma, come dicevo prima e come è di solare comunicata evidenza, il «silenzio assordante» che il Presidente del Consiglio (che non è il tutore dei suoi Ministri, anche se invero a volte sembra che la detta funzione una sua ragion d'essere l'avrebbe pure, ma che è tuttavia il responsabile politico di quanto essi fanno e dicono), si è dapprima riservato, per poi calarsi nel precipizio di una delle sue proverbiali banalità, cui, per la verità, ci ha da sempre abituato nelle sue apparizioni televisive: «Il Governo rispetta l'assoluta indipendenza della Corte».

l'opinione dell'onorevole Pecoraro Scanio non è certo quella del Governo; e ancora: «chi è il sottosegretario Naccarato?». Ma sarebbe stato probabilmente troppo chiedere. Dunque, la questione è quella dell'«assordante silenzio», dapprima, e del «vuoto spinto», poi, in relazione alla convinzione, pubblicamente comunicata da Ministri, che la Corte costituzionale, l'istituzione posta ad essere la massima custode della nostra democrazia, fosse in realtà disponibile «per tutte le stagioni», che i suoi giudici siano in realtà marionette disponibili per i *desiderata* della politica di turno. E tutto ciò, per non voler cadere nella suggestione delle parole non dette, di una Corte «amica» del Governo in carica, perché formata da giudici di sinistra o comunque indicati dalla sinistra. Non perderò tempo, signor Presidente, né farò perdere tempo ai colleghi nell'Aula e al signor Vice presidente del Consiglio nello stare a dire qui della rozzezza, dell'inopportunità, della pericolosa deriva antidemocratica - perché di questo si tratta - che è nelle parole che i componenti del Governo, che oggi hanno scomodato a loro improbabile difesa proprio l'onorevole Rutelli, hanno consegnato al dibattito politico e hanno fatto registrare dalla stampa. Voglio viceversa parlare di altra loro decisiva «non qualità». E mi voglio rivolgere, signor Presidente, a lei ovviamente (per debito e costume di questa Camera), ma anche direttamente non solo all'onorevole Rutelli, che qui oggi rappresenta il Governo, pure e soprattutto ai *leader* delle forze politiche che questo Governo hanno determinato e che a questo Governo assicurano ripetute fiducie e quindi vita permanente. La decisiva «non qualità» dei componenti di questo Governo, che sono chiamati oggi in causa, è quella della loro totale inadeguatezza rispetto all'esigenza che essi siano Ministri di tutti i cittadini, che essi siano rappresentanti opportuni (in Italia, in Europa e in ogni altro consesso internazionale) di nevralgici centri d'interesse e di regolazione di diritti nel Paese. È a costoro È a costoro consentita, signor Vice presidente del Consiglio, sul piano personale, la rozzezza, la banalità, la presuntuosità, ma non è loro consentita, nella loro veste pubblica, l'inadeguatezza di una condotta che è determinativa di ragione di discredito, di perdita di fiducia rispetto ai cittadini, di un'istituzione in cui gli stessi hanno diritto di credere come ultimo baluardo dei loro diritti e non certo, come vorrebbero i predetti «uomini di Governo», come ultimo baluardo dei rispettivi appetiti antireferendari, a tutela della resistibilità della politica piccola piccola di cui sono portatori e nemmeno sani. Signor Vice presidente del Consiglio, «questi uomini di Governo» vanno dimessi dal Governo e della questione non parliamo più. È successo per molto meno in altre democrazie; ci faccia credere che può succedere anche qui e rinunci - come invece ha inteso fare - ad invocare l'assoluzione di condotte che sono state inammissibili (inammissibili e basta) richiamandosi alla pronuncia con cui la Corte costituzionale si è espressa sulla vicenda. La Corte - come lei ha ricordato - ha ribadito che è nella sua collegialità la propria indipendenza ed autonomia. E che doveva dire la Corte? Che non è così? Che l'acqua calda non è calda? Tale suo approccio, in verità, signor Vice presidente del Consiglio (mi spiace dirlo), è in realtà solo proporzionato con l'abituale, anche sua di oggi, invocazione conclusiva, secondo cui "è necessario abbassare i toni da parte di tutti": ovviamente e generosamente. Quasi quasi, sembra, signor Vice presidente del Consiglio, al termometro delle banalità, che lei qui oggi abbia letto un intervento di vero e proprio pugno del presidente Prodi.

l'età in cui il carattere può prevalere sulla ragione, onde per cui eviterò - per così dire - di abboccare all'amo propagandistico lanciatomi dalla senatrice Palermi. Il tempo a disposizione è poco, ma ne potrei rubare una frazione per ricordare alla senatrice Palermi come quel testimone fidefacente, l'onorevole Mancuso, sia esattamente quel parlamentare che il centro‑sinistra ostinatamente non ha voluto alla Corte costituzionale, salvo poi - proprio in ragione di quelle dichiarazioni - applaudirlo ogni volta che interveniva. E ancora, senatrice Palermi, mi consenta è difficile che il centro-destra possa aver criticato la Corte costituzionale per la pronuncia sulla legge ex Cirielli, in quanto - come lei dovrebbe sapere - il senso di quella stessa pronuncia era che la disciplina sulla prescrizione era troppo restrittiva, poiché non si allargava anche ai procedimenti in primo grado: questo solo per onore di verità. di verità. Signor Vice presidente del Consiglio, credo che lei sia venuto qui a rispondere in maniera molto burocratica ad un problema estremamente grave e non inusuale o serio, come ella ha ritenuto di doverlo definire. Quello che qui è in discussione è il rapporto che deve sussistere fra i vari organi dello Stato e, in particolare - se si vuole - tra l'Esecutivo e il supremo organo di garanzia della nostra Costituzione, per l'appunto la Corte costituzionale. Vede, signor Vice presidente del Consiglio, indipendentemente da quanto pure è stato affermato, sempre - credo - dalla senatrice Palermi, cioè che ciascuno può esprimere le opinioni che meglio ritiene anche con riferimento alla Corte costituzionale, mi permetto di ricordare a lei, alla stessa senatrice e ai colleghi senatori quanto ha affermato il Presidente della Repubblica: quando un problema è portato di fronte alla Corte, non se ne deve più discutere. Tanto meno ne devono discutere le persone che, in ragione del loro ruolo governativo e delle loro *leadership* politiche,

che le persone che - secondo la stampa - sono state, per così dire, verbalmente più entusiaste in riferimento alla decisione della Corte sul *referendum* siano per l'appunto i *leader* di quei partiti che da un certo esito referendario trarrebbero i maggiori danni. Vede, signor Vice presidente del Consiglio,

per rispetto all'autonomia e all'indipendenza della Corte, (e lasciamo perdere la *boutade* sulla divisione dei poteri, sulla quale già si è soffermato il senatore D'Onofrio). Ma qui sono proprio l'autonomia e l'indipendenza della Corte a essere in discussione. Almeno in questa sede,

un Sottosegretario di Stato (mi pare fosse un Sottosegretario al Ministero dell'interno) ebbe un'accesa formulazione verbale nei confronti di un potere dello Stato: il centro-sinistra insorse e quel Sottosegretario si dimise. Non vedo, non sento, non registro nulla che riguardi le eventuali dimissioni del sottosegretario Naccarato ovvero del Ministro dell'ambiente. dell'ambiente. Nel caso del sottosegretario Naccarato, poi, non si tratta di una frase aggressiva, ma di un'accusa specifica d'interferenza, rivolta al Presidente della Repubblica nei confronti della Corte costituzionale; si tratta, per essere chiari, dell'accettazione di questa interferenza specifica da parte della Corte costituzionale. Senatrice Boccia, sulle dimissioni non c'è nulla di intrasparente o di strumentale. Le dimissioni si danno, in genere sono respinte e, in genere, non si reiterano. Nel caso di specie, invece, vengono reiterate. Se il senatore Storace mi consente di mutuare e di adattare al caso di specie una frase a lui cara, potrei dire che se un uomo non è capace di dimettersi irrevocabilmente per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non valgono niente le sue dimissioni. Su questo, magari, potete fare un approfondimento

forse voi non avete fatto attenzione al provvedimento della Corte costituzionale, la quale - badate bene - ha affermato che quelle dichiarazioni vi erano state,

reso non proprio il dire del Ministro dell'ambiente o del Sottosegretario di Stato. Davvero devo dire: è un prendere le distanze affermare che si è rispettosi dell'autonomia e dell'indipendenza della Corte costituzionale o è solo un'ovvietà?

Credo, signor Presidente, signor Vice presidente del Consiglio e signori del Senato, che il Governo abbia perso una grande occasione per cercare di fare chiarezza su un episodio gravissimo; un episodio che per l'ennesima volta non individuerà gli autori di un misfatto istituzionale, vale a dire di una pressione inaudita e gravissima nei confronti della Corte costituzionale; mi viene da ricordare a chi afferma che con voi è arrivata la serietà al Governo, che la serietà è cosa diversa dalla tristezza, ma che tra l'essere triste e l'essere tristo, come il Griso di Manzoni, ne passa poco e che, nel caso di specie, essendo i bravi che hanno aggredito la Corte ancora in servizio, probabilmente invece che triste sarebbe meglio chiamarlo tristo.

desidero ringraziare il Governo per la sobria e puntuale ricostruzione dei fatti, per il comportamento tenuto nel corso della vicenda che ci occupa ed in particolare per la posizione chiara e netta assunta tempestivamente dal Presidente del Consiglio. Tra i valori fondanti per una democrazia vi è senz'altro la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tutti siamo chiamati al rispetto di questo principio cardine del nostro sistema istituzionale, in primo luogo coloro che esercitano funzioni pubbliche. E quando è in questione la suprema magistratura, il giudice delle leggi, il principio si fa ancora più cogente. Anche un certo riserbo sarebbe opportuno, ma dinanzi alla richiesta di aprire un dibattito parlamentare non ci si può trincerare dietro queste considerazioni, ma va affrontato il tema e colta l'occasione per rimarcare i profili di fatto di una vicenda sicuramente eccezionale, per alcuni versi singolare, e per cercare di condividere alcune osservazioni sui confini entro i quali ciascuno è chiamato a svolgere le proprie funzioni. Voglio dire subito (ma non per aprire una polemica, perché sarebbe eccessivo da parte mia ed anche perché il contenuto di questo mio intervento, come vedrete presto, sarà in tutt'altra direzione) che noi, nel momento in cui celebriamo il rispetto sommo dovuto alla Corte costituzionale, che è il giudice delle leggi, il garante della Costituzione, dovremmo - mi rivolgo al collega Palma garantire la stessa osservanza nei confronti della Presidenza della Repubblica, non soltanto di quella in carica, ma anche di quella del presidente Scalfaro, che è stato inflessibile e rigoroso tutore della nostra Carta costituzionale. Non voglio semplificare la questione, non voglio riportarla nell'ambito del rapporto tra Governo e Corte costituzionale, tra politica e magistratura. Condivido le osservazioni, come sempre acute, del collega D'Onofrio sulla questione che involge strettamente il campo e la sfera della politica, ma non c'è dubbio che nella questione delle dimissioni del professor avvocato Romano Vaccarella ci siano dei profili più complessi, che meritano alcune considerazioni. Come sempre, come in tutte le vicende umane, alcuni di questi argomenti sono chiari fin d'ora, li stiamo discutendo; altri, come al solito, li conosceremo più avanti nel tempo.

debba essere invocato il silenzio dei politici contro ogni interferenza nei confronti della Corte quando si tratti di materie che riguardano - come ha detto il collega D'Onofrio - così significativamente la sfera della politica. Stiamo parlando della legge elettorale*,* stiamo parlando di *referendum* per i quali la raccolta delle firme è appena cominciata e questo silenzio sarebbe ancora più singolare, posto che - replico brevemente al collega Palma - non è ancora detto che la Corte mai si occuperà di questa vicenda. Concordo sul fatto che, una volta rimessa la questione dinanzi alla Corte costituzionale, sarebbe opportuno un più rigoroso riserbo, ma le firme debbono essere ancora raccolte, il Senato si sta occupando della vicenda e qui invece stiamo sostenendo che tutti noi dovremmo tacere. Abbiamo, però, anche

fermo restando il rispetto dell'istituzione e soprattutto il rispetto delle sue decisioni. Vi debbo dire con franchezza che, se le motivazioni della decisione del professor Vaccarella di dimettersi irrevocabilmente da giudice della Corte, dopo cinque anni e quattro giorni dal suo insediamento, stanno davvero nelle dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo a proposito dell'ammissibilità dei quesiti referendari sulla legge elettorale, la scelta mi sembra davvero eccessiva e poco comprensibile. E non potrà non riflettere lo stesso interessato, insieme a noi, come tra qualche giorno nessuno si ricorderà più delle motivazioni delle sue dimissioni, ma tutti si ricorderanno del fatto che si è dimesso, avvenimento che sostanzialmente non ha precedenti nella storia della Corte costituzionale. Dice la Corte che la maggior tutela della sua indipendenza è nella collegialità delle sue decisioni. Mi chiedo e chiedo a voi: è possibile che il professor Vaccarella non si sia reso conto del fatto che, violando quella collegialità, abbia danneggiato proprio quell'indipendenza che gli stessi giudici della Corte hanno rimarcato unanimemente nel respingere e nell'accettare poi le sue dimissioni? E non si è posto il problema di quanto queste dimissioni possano interferire - sono certo senza successo - sulle decisioni future, se ci saranno, della Corte costituzionale? Lo stesso collega Saro, con la sua limpida onestà intellettuale, ha detto - come riportato nei resoconti stenografici di oggi - che probabilmente la Corte, se mai sarà chiamata a pronunciarsi, un'ammissibilità la concederà perché sono intervenute le dimissioni del professor Vaccarella. Non intendo dare consigli al professor Vaccarella, ma auspicavo un ripensamento e la sua adesione alla richiesta formulata congiuntamente da lei, signor Presidente del Senato, e dal Presidente della Camera. L'avere insistito, sostenendo generiche le assicurazioni del Presidente del Consiglio, non mi ha convinto e credo non abbia convinto molti altri, che attendono di conoscere se vi sono ulteriori motivazioni rispetto a quelle che sono state riportate nella lettera di dimissioni presentata, non solo al Presidente della Corte, ma irritualmente ai Presidenti delle Assemblee parlamentari e al Presidente del Consiglio. Per di più, rimane del tutto in comprensibile - lo dico con chiarezza - il suo dolersi del silenzio istituzionale in difesa delle prerogative della Corte, posto che sono intervenute tutte le più alte cariche dello Stato: Stato: il Presidente della Repubblica, invitando tutti al rispetto della Corte, il Presidente del Consiglio, per assicurare l'impegno del Governo a difesa del principio, ed anche congiuntamente - come ho detto - i Presidenti di Camera e Senato, che lo invitavano a ritirare le dimissioni e la stessa Corte, che ha respinto unanimemente e con un argomentato provvedimento le sue dimissioni. Non ho capito e non riesco davvero a comprendere chi altri sarebbe potuto o dovuto intervenire. Ribadisco, ancora oggi, che si tratta di una questione della quale la Corte dev'essere ancora formalmente investita. Non intendo eludere il tema posto all'attenzione dal professor Vaccarella, cioè le opinioni espresse da alcuni esponenti del Governo in merito all'ammissibilità dei quesiti referendari, né intendo aprire una polemica tra maggioranza e opposizione in questa materia, ma trovo assai più grave censurare le sentenze della Corte, come ha fatto il presidente Berlusconi il 24 gennaio scorso quando, dinanzi alla dichiarazione di illegittimità della legge Pecorella da parte della Corte, dichiarava che non c'è democrazia, o come nel caso del conflitto di attribuzioni che riguardava l'onorevole Bondi, il quale il 9 marzo scorso su una questione che lo riguardava direttamente affermava dopo la sentenza: «Ringrazio i giudici della Corte costituzionale per avermi ricordato che viviamo in un Paese incivile». Ma l'offesa più grave alla Corte, il più micidiale atto di delegittimazione - se me lo consentite - sta proprio nelle parole di questi giorni del presidente Berlusconi, il quale svolge un calcolo sulla collocazione politica dei giudici della Corte fissandolo in un 11 a 4 a suo sfavore, un po' come il risultato delle ultime elezioni regionali. Anch'io il 26 aprile del 2002 ho votato il professor Vaccarella quale giudice della Corte costituzionale, ed ero certo, e sono sempre stato certo in questi cinque anni e quattro giorni del suo mandato, che avrebbe dato un contributo formidabile, con la sua competenza professionale e il suo equilibrio, al lavoro della Corte costituzionale; non ho mai pensato che fosse un esponente della destra di questo Paese. I giudici della Corte sono giudici, cari colleghi, e a nulla vale la loro provenienza. Non è un gioco di casacche. Il giorno dopo l'assunzione delle loro funzioni la loro fedeltà è solo nei confronti delle istituzioni che sono chiamati a servire, ed il loro principale dovere è assicurare la piena imparzialità. Eppure, nonostante queste gravissime dichiarazioni, la suscettibilità del professor Vaccarella non ne è uscita scossa, né sono intervenute dimissioni di alcun genere. Sono convinto che le istituzioni giudiziarie si difendono principalmente con la qualità dei provvedimenti che vengono emanati e la migliore tutela, come saggiamente ha detto la Corte, sta proprio nella collegialità dell'organo e nell'evitare ogni personalismo. Non è rilevante il merito, ma vale la pena di sottolineare che la materia dell'ammissibilità o meno dei quesiti referendari appartiene ad una giurisprudenza assai vasta della Corte, anche per l'uso non sempre proprio che nel tempo si è fatto di questo importantissimo e delicatissimo strumento. Tanto è ricca la casistica, tanto sono chiari i princìpi che sono stati espressi. Al supremo organo della giustizia costituzionale ci affidiamo interamente, ma credo che nessuno debba perdere il diritto a discutere, anche nel merito, di un avvenimento non trascurabile della vicenda politica del nostro Paese, nel dovuto rispetto delle istituzioni, della Corte costituzionale, della sua decisione e soprattutto perché la Corte solo fra sette mesi probabilmente sarà chiamata ad occuparsene. Né mi sembrano da accogliere le proposte di deroghe ed eccezioni, ritenute ammissibili dal professor Vaccarella, per cui ne possono parlare solo gli esponenti politici che siano titolari anche di incarichi accademici. Da questa vicenda, sproporzionatamente a mio avviso drammatizzata, non dobbiamo trarre conclusioni semplicistiche e soprattutto non dobbiamo consentire che il tema della difesa delle nostre istituzioni

da quelle per le quali il confronto di diverse posizioni non è solo opportuno, ma addirittura una ricchezza per la nostra democrazia. Fortunatamente, in questo senso la stessa Costituzione ci offre un immediato monito ed un richiamo alla maggiore convergenza della politica in materia istituzionale, poiché tra pochi giorni saremo chiamati, insieme, cari colleghi, ad eleggere un nuovo giudice della Corte costituzionale in sostituzione del professor Vaccarella. Ed insieme sono certo che, con buona volontà, troveremo la personalità più adatta a confermare l'enorme prestigio, anche internazionale, della nostra Corte costituzionale e a proseguire questo lavoro ininterrotto che dal 1956 illustra la Corte, grazie alla modernità della nostra Carta costituzionale, come un formidabile strumento per il progresso democratico della nostra Nazione. *(Applausi

fa proprio il documento XXII, n. 14, relativo alla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

atti dell'Assemblea costituente alla mano, che, quando l'Assemblea dovette decidere sulle materie per cui non era ammesso il *referendum*, aveva il testo della Commissione dei 75 che faceva riferimento trattati internazionali, amnistie e condoni e materia tributaria. In Aula, da parte di una costituente

certo, la forma conta, ma la sostanza era che l'Assemblea costituente aveva voluto escludere le leggi elettorali dai*referendum*.